Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» (1819). Il provvedimento è stato assegnato in data odierna alla Commissione affari costituzionali per i presupposti di costituzionalità, nonché alla Commissione bilancio per l'esame in sede referente, con i pareri di tutte le altre Commissioni permanenti che dovranno essere espressi alla Commissione di merito entro otto giorni da oggi.

Oggi pomeriggio si passerà immediatamente al seguito della discussione dell'assestamento del bilancio dello Stato, a conclusione della quale saranno effettuate le votazioni finali - con la presenza del numero legale - dell'assestamento medesimo e del rendiconto. Si passerà poi all'eventuale seguito del disegno di legge sullo sportello unico delle imprese. Domani mattina, dopo l'esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia, si passerà alla discussione delle mozioni su Alitalia-Malpensa, per le quali sono stati ripartiti tempi tra i Gruppi. Nel pomeriggio di domani, con inizio alle ore 16, saranno discusse le mozioni sul vice ministro Visco, anche in questo caso con ripartizione dei tempi. Nella seduta antimeridiana di giovedì 4 ottobre sarà esaminata la Nota di aggiornamento al DPEF, sempre con ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nel pomeriggio di giovedì il Presidente renderà comunicazioni sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Avrà quindi inizio la sessione di bilancio: le Commissioni in sede consultiva trasmetteranno i propri rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 17 di lunedì 15 ottobre; la 5a Commissione permanente concluderà l'esame dei documenti finanziari entro martedì 30 ottobre. La prossima settimana, salvo che argomenti urgenti non lo richiedano, l'Assemblea non terrà seduta per consentire il lavoro delle Commissioni sui documenti finanziari. Nella settimana successiva alla prossima, l'Assemblea si riunirà nelle giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18 ottobre per l'esame del decreto-legge sull'avvio dell'anno scolastico, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati e concluso dalla Commissione competente, nonché per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi. Nel corso di tale settimana la Conferenza dei Capigruppo definirà gli ulteriori tempi della sessione di bilancio.

giovedì, tra i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria ve ne è uno che traduce in atto normativo l'accordo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali.

del 27 settembre sono stati votati gli ordini del giorno G1, G2 e G3. Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana del 26 settembre ha avuto luogo la votazione degli articoli del rendiconto.

Chiedo, signor Presidente, che il Governo risponda puntualmente sulla questione. Il Governo, nel corso dei mesi passati, attraverso l'emersione di cinque tesoretti successivi, più il sesto, quello di mercoledì della scorsa settimana, è arrivato a dire formalmente che le entrate complessive delle pubbliche amministrazioni per l'anno in corso ammontano a circa 727-728 miliardi di euro, contro i 703 miliardi di euro che Governo e Parlamento avevano votato a dicembre. Ricordo, signor Presidente, che questo è l'unico atto formale in corso d'anno con il quale si va a modificare il totale del gettito, da 703 miliardi alla cifra emersa in corso d'anno. allora, due questioni. Anzitutto, come mai il Governo, avendo dichiarato circa 729 miliardi di gettito complessivo per l'anno in corso 2007, nella Nota di aggiornamento al DPEF prevede soltanto 722 miliardi? Che fine hanno fatto i sette miliardi dichiarati dallo stesso Governo? Come mai non sono stati correttamente inseriti nella Nota di aggiornamento? Inoltre, di quei 722 722 miliardi scritti nella Nota di aggiornamento al DPEF pubblicata ieri dal Governo, come mai nel bilancio di assestamento che stiamo discutendo in questo momento l'incremento di gettito pari ai 25 miliardi dichiarati dal Governo, inserito nella Nota di aggiornamento al DPEF per soli 19 miliardi in più, nel bilancio di assestamento in esame, diventa soltanto di 12,9 miliardi? In merito, signor Presidente, è necessario che il Governo dia una risposta chiara e trasparente, facendo luce su un duplice mistero. In primo luogo, perché il gettito dichiarato dal Governo attraverso sei successivi tesoretti (che, continuo a sostenere, rappresentano la controprova dell'approvazione a dicembre di una posta di bilancio falsa), quei 25 miliardi in più dichiarati dal Governo, diventano

nella Nota di aggiornamento al DPEF comunicata ieri al Parlamento, sulla base della palese sottostima che ancora nasconde sette od otto miliardi di gettito per l'anno in corso,

coerentemente con la sottostima del 2007, ma che nasconde sul 2008 almeno 10 miliardi di gettito tendenziale. Ebbene, questo inficerà tutta la discussione che svolgeremo in Parlamento sulla prossima legge finanziaria.

ancora occultato in questo momento; inoltre, risulterà che tutta la finanziaria per il 2008 è basata su un andamento tendenziale di gettito che oggi il Governo ha indicato

Il Governo - se durerà - nel corso del 2008 prepara ancora la scoperta di ulteriori tesoretti dovuti e assegnabili alla sua pervicace lotta all'evasione; invece, i dati emersi ieri dimostrano che fino a oggi non c'è un euro in più di lotta all'evasione, ma 25 miliardi di gettito occultati. Di questi, il Governo ne fa emergere 19 nella Nota di aggiornamento al DPEF e soltanto 12 nell'assestamento di bilancio che stiamo discutendo. Signor Presidente, la prego di chiedere che il Governo risponda su questo, non soltanto e semplicemente all'opposizione, ma soprattutto alla sua maggioranza, perché sta nascondendo alla sua maggioranza l'andamento vero del gettito, che porta, peraltro, a partire dai dati consuntivi del 2006, nel corso del 2007 e del 2008, ad alcuni risultati. Concludo con l'ultimo dei misteri, signor Presidente, e vorrei che i colleghi della maggioranza

perché con la spesa che il Governo ha già deciso il *deficit* di quest'anno raddoppia al 2,4 per cento e le spese dell'anno prossimo sono già predeterminate, indipendentemente dai voleri, dalle richieste e dalle esigenze anche delle singole componenti di questa maggioranza di Governo. Quindi, il mistero è che se ci sono più entrate ci deve essere meno *deficit*, oppure il Governo dica chiaramente che ci sono più spese e che quelle per il 2008 saranno molte di più di quelle che ha indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nella Relazione previsionale e programmatica di quest'anno. Non è infatti possibile che con un andamento *record* del gettito, che porta la pressione fiscale dal 40,6 di fine 2005 al 43,1 (dati ufficiali del Governo), il *deficit* non solo non si riduca, ma aumenti rispetto agli andamenti tendenziali. Colleghi della maggioranza, siete consapevoli che quando vi dicono che non c'è più un euro per ciascuna delle vostre richieste ciò corrisponde ma semplicemente perché il Governo vi ha nascosto le entrate e continua a nascondervi gli andamenti della spesa, decisi nel chiuso di dodici o tredici Ministeri e non in trasparenza nelle Aule parlamentari? *(Applausi dai Gruppi AN e

tiene conto dell'andamento effettivo del gettito nei primi otto mesi dell'anno. Ricordo che, allorché è stato presentato il disegno di legge di assestamento a giugno, i dati previsivi si fondavano prevalentemente sugli scenari macroeconomici che erano fino a quel momento noti e non potevano minimamente tener conto dell'andamento effettivo degli incassi relativi all'imposta autoliquidata, in quanto gli stessi vengono riscossi a partire dal mese di luglio. Il principale oggetto dell'emendamento, quindi, di queste maggiori entrate, che inizialmente erano state stimate in circa 5 miliardi di euro e che successivamente sono state elevate di ulteriori 900 milioni, con l'ultimo emendamento presentato la scorsa settimana. Queste maggiori entrate possono essere fondamentalmente ricondotte a due componenti. La prima, che ha portato a maggiori introiti IVA e a minori introiti per imposte dirette, riguarda un diverso andamento del gettito relativo alla cosiddetta sentenza «IVA auto». In altre parole i contribuenti, forse per un periodo iniziale di incertezza, non si sono avvalsi, come inizialmente atteso, della facoltà di dedurre pienamente le spese relative all'acquisto di nuovi autoveicoli ad uso professionale. Questo ha comportato, con segno diverso, variazioni nei tributi IVA, IRE e IRES. Dall'altro lato va, invece, sottolineato un buon andamento delle altre imposte dirette, in particolare di quelle autoliquidate, che denotano il favorevole andamento dell'economia. Ricordo per memoria che l'imposta autoliquidata si riferisce, per la parte del saldo, agli imponibili relativi all'anno precedente, quindi al 2006, e, per quel che riguarda l'acconto, agli andamenti in atto.

alle attese. In parte ciò è anche riconducibile ad un periodo invernale relativamente mite, che ha determinato un minore consumo di combustibile. Per quanto attiene alle spese, al di là di alcune compensazioni e diverse allocazioni che sono state chieste dai Ministri di settore, al fine di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'azione dei Ministeri da loro diretti,

i contributi al finanziamento del bilancio comunitario, in quanto è stato comunicato con certezza quanto è l'ammontare dovuto dall'Italia per l'anno in corso (e questo ammontare è nettamente inferiore, di oltre un miliardo, a quanto era stato inizialmente accantonato per provvedere agli obblighi comunitari); dall'altro lato, vi sono variazioni di importo meno rilevante,

nei confronti dell'azienda di radiodiffusione) e una rideterminazione degli esborsi per le vincite al lotto, che recepisce un andamento meno favorevole del previsto delle giocate stesse. Per sommi capi, questa è la descrizione del contenuto dell'emendamento. Sottolineo che la parte prevalente e la parte positiva riguardano questo favorevole andamento delle entrate, del quale si è avuto modo di

presentazione della finanziaria avvenuta - come il sottosegretario Sartor certamente saprà - davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato qualche giorno fa, parla di un altro Paese, non del nostro. Gli spostamenti evidenti sul fronte dei risultati di maggiore pressione fiscale a carico delle famiglie, delle imprese, del lavoro

rappresentanti del Governo, continuate però a far sparire in quel pozzo nero di maggiore spesa pubblica, che solo manipolando i dati potete poi dire di aver ridotto.

Sennonché, l'obiettivo era quello di spremere gli italiani di ulteriori tasse: e voi ci siete riusciti all'inverosimile! E per cosa avete fatto

a tirare a campare, o a far campare, il Governo Prodi, cioè il Governo con il più basso gradimento popolare nella storia di questo Paese; a migliorare, non la qualità dei servizi offerti ai nostri cittadini con i soldi pubblici, ma ad aumentare le strutture, che qualche volta sono buone ma molto più spesso non lo sono in quanto inefficienti, spesso antidiluviane, ancor più spesso contrarie e ostili ai cittadini.

Quale effetto avete ottenuto? Di sicuro, quello di aver depresso la nostra economia proprio mentre gli altri Paesi della zona euro, pur con difficoltà, guadagnano qualche punto in termini di produttività e di formazione del Prodotto interno lordo; di mortificare, soprattutto, la voglia degli italiani di lavorare e di intraprendere, caricandoli all'inverosimile di tasse senza nessuna forma di rispetto per quel denaro pubblico che, invece, dovremmo trattare con maggiore parsimonia. Proprio a questo mirano gli emendamenti da noi presentati, e che vado velocemente ad illustrare. Essi mirano, fondamentalmente, a contenere quella spesa o, almeno, a razionalizzarla, laddove

versa. Per esempio, a proposito degli interessi sui titoli del debito pubblico il Governo riesce a fornire dei numeri e delle previsioni e ad assestare questo bilancio non tenendo conto di quanto avviene non solo nel Paese, dove

una variazione in aumento di 100 milioni di euro per un settore che, già pesantemente colpito dal decreto Bersani dello scorso luglio, ha visto ridurre pesantemente lo stanziamento pubblico al Ministero, che invece a

spero con un po' di tempo a disposizione, sulla tabella dello stato di previsione del Ministero della giustizia, sulla voce Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

il minimo importo utile a tentare di affrontare una profonda crisi che, nonostante l'indulto (che tanto è costato a questo Paese ed anche alla coscienza di questo Parlamento), noi affrontiamo di nuovo in termini di emergenza per l'affollamento della carceri. I dati più recenti mostrano che le carceri sono già vicine al limite massimo di capienza, se mi è consentito l'utilizzo di questo brutto termine, visto che parliamo di esseri umani,

per non essere costretti a ripetere, tra qualche anno, un indulto che ha seminato molto sconcerto nel Paese. Non serve che mi dilunghi su questo argomento. Sono certa che la sensibilità di tutti faciliti la comprensione su quanto questo atto sia

e soprattutto utilizzi ancor più frequentemente i mezzi d'informazione pubblici o privati per far passare un concetto che poi viene smentito nella realtà delle cose, per cui

un po' comica, perché parlare di autorevolezza a proposito del ministro Pecoraro Scanio è - ahimè - cosa un po' ridicola, visto che viene smentito a ogni piè sospinto dai più grandi scienziati e dai tecnici davvero competenti in materia di politiche ambientali. Noi vi chiediamo comunque di apportare questa variazione per dare il segno di una maggiore attenzione che tutti noi dobbiamo avere e dobbiamo continuare a far crescere rispetto all'ambiente, dove il piano energetico nazionale costituisce una delle colonne portanti del tipo di ambiente e di mondo che noi vogliamo costruire.

sembra infatti che la questione dei mezzi operativi e strumentali del Ministero dell'interno e quindi delle Forze di polizia, scritta così possa sembrare solo una questione tecnica, tradotta nella realtà vuol dire che spesso - come sappiamo - le nostre questure, i nostri poliziotti non hanno le macchine per poter uscire e compiere il loro servizio, o spesso quelle autovetture oltre i 200.000 chilometri, si sa, sono sfinite, ma non abbiamo i soldi per sostituirle, quindi per mettere a disposizione delle Forze di polizia mezzi operativi sul serio efficienti. Per non parlare poi dell'emergenza incendi, che anche quest'anno ha messo a nudo...

stabilire, ristabilire e sottolineare in questa sede quella differenza che è stata fatta anche oggi e in questi giorni. Presidente, scusi, mi consente di poter cambiare postazione per parlare?

di capire e discernere i fatti della politica e dare qualche chiarimento a chi ci domanda cosa succedendo e in principal modo quando cadrà il Governo - nel fondo di Sartori c'era una acuta dissertazione che stabiliva con riferimento semantico alla differenza tra democrazia e demagogia, perché tutte e due le parole

...alla decisione popolare l'indirizzo sull'azione di amministrazione e di governo, invece demagogia è cercare

guardi che in quest'Aula probabilmente non parleremo di finanziaria, perché, per quanto si dica che dobbiamo discutere la finanziaria votando tutti gli emendamenti e tutti gli articoli, visto che questi stanno lievitando velocemente, così come avevamo previsto, da 100 a 126, poi c'è il collegato di sessione e il decreto e quindi si tratterà di una baraonda che sarà molto vicina ai 1.700 commi della finanziaria passata, l'unico modo per parlare un po' di economia è rappresentato da quelle fasi che precedono la trattazione della finanziaria, perché poi probabilmente ne parleremo soltanto in Commissione. Ora, il punto sostanziale è quello di vedere come arrivano questi soldi, perché l'impegno che avevamo preso

non soltanto il modo sommesso con cui Governo è venuto a dirci da dove vengono gli ulteriori 900 milioni di euro: di questo stesso tono è stato l'intervento in Commissione, in cui si è trattato di 5 miliardi di euro. E lo stesso tono è stato usato quando ci ha detto come si stanno spendendo

è l'esito di un'azione demagogica del Governo; come diceva il senatore Baldassarri, il Governo ci dice che entrano i soldi soltanto nel momento in cui ha già deciso come spenderli, e non lo dice mai

la distrazione del Governo e la distrazione della Presidenza, perché la volontà ultima è quella di fare assolutamente l'assestamento. Il fatto che l'assestamento si stia facendo in ritardo signor Presidente, non è colpa nostra.

in canali di richiesta partitica o politica o per prebende a questo o a quell'altro soggetto - ma per dire la verità rispetto a certi capitoli di bilancio. Oggi si dice che nella finanziaria verranno implementate e incrementate le risorse per le Ferrovie e per l' ANAS, quando questa era stata una delle critiche fatte al vecchio Governo dal nuovo Governo, che aveva sostenuto di aver trovato un buco perché nel bilancio

le opere e la definizione di opere già fatte. Contemporaneamente però sappiamo che le Ferrovie sostengono di non avere le risorse necessarie per poterle completare. E allora noi presentiamo un emendamento per trasferire

con il significato di un altro emendamento che abbiamo presentato. Il Governo ha fatto uscire completamente dall'agenda la necessità di trasferire risorse per il Meridione,

vituperabile ed esecrabile demagogia, dice tutto e il contrario e di tutto all'interno della stessa compagine. E allora quello che chiediamo con un nostro emendamento è che ad esempio vengano implementati i fondi del FAS

dopodiché abbiamo visto che questi soldi erano nettamente inferiori a quelli dell'anno passato, ma non soltanto: vediamo che quei fondi non sono stati utilizzati per il Meridione, per cui nulla è stato fatto, ma sono stati utilizzati oggi per la copertura del decreto e allora come fare a non parlare in quest'Aula della necessità di implementare le risorse per il FAS? Lei, signor Presidente, forse non saprà, come non sanno molti colleghi, che il decreto interministeriale della fine di luglio per la ripartizione delle somme finalizzate ad onorare le richieste, per cui si era costruito un certo diritto legittimo, del prestito d'onore,

il decreto interministeriale non è stato fatto bene. Nell'uno e nell'altro caso, abbiamo superato la fine di settembre, anzi è già iniziato il mese di ottobre, la ripartizione dei fondi è stata fatta a luglio e il prestito d'onore non prevede che ci sia la possibilità, allo stato dell'arte, che i soldi arrivino in tempo per quelli che ne avevano fatto domanda. Allora cosa stiamo chiedendo di più, signor Presidente? Di parlare della necessità di implementare questi fondi: come si può non occuparsi di aree sottosviluppate, di ferrovie? E poi altro emendamento di cui parlare. Oggi sentiamo dire da tutti i giornali che una delle previsioni fatte è quella per onorare gli impegni stipulati in sede comunitaria per l'«Eurofighter» e quella per le fregate italo-francesi della classe FREMM; non si capisce come i soldi che erano stati resi disponibili nelle finanziarie 2003 e 2004 non siano stati spesi nel 2006 e ci sia la necessità oggi di implementarli con la finanziaria dell'anno prossimo. Perché non farlo con l'assestamento? Perché prevedere che i 9 miliardi che derivano dagli emendamenti presentati all'assestamento debbano essere spesi con il decreto, con una fiducia e contemporaneamente alla finanziaria senza che abbiamo la possibilità di discuterne all'interno dell'assestamento?

ulteriormente di questo problema, che è a nostro parere un problema di grandissima importanza, la ringrazio del tempo che mi ha concesso.

forse unica di poter arrivare al Governo, al di là dei numeri, e di poter impostare una politica economica più avanzata, che non fosse quella del giorno dopo,

perché anche voi, purtroppo, non riuscite ad andare al di là del contingente, del domani, e allora per tamponare le richieste che arrivano oggi da Grillo, domani dai compagni della FIOM, dopodomani dai disubbidienti di Vicenza ed il giorno prima da qualche altro portatore d'interesse, la barca non si riesce più a tenere. Allora, Presidente, arrivano gli assestamenti, i tesoretti, la speranza che con questo tesoretto si possa trovare finalmente la colla che possa tenere assieme una maggioranza che va dal Sud Tirolo, che è molto preoccupato per le proprie funivie, al collega dei Verdi, che è molto preoccupato dal creare le premesse per il prossimo *blackout* (che avremo sicuramente, perché i rigassificatori non ci sono più), al collega Loiero, che deve assumere qualche migliaia di di forestali e che grida: «Grande vittoria, il Governo mi ha promesso che ne assumeremo anche qualche migliaio!». Ma che vittoria e vittoria! Questa è una sconfitta per tutti, anche per i calabresi. Quindi,

Avevano ragione i colleghi che mi hanno preceduto nel dire come la manovra politica concreta sia quella di tenere bassi i numeri e poi tirarne fuori altri all'ultimo momento, e lo ripeteremo; questi 900 milioni di euro sono arrivati

«È arrivato un altro tesoretto», 900 milioni di euro che sono andati: tre milioni alla senatrice Montalcini; qualche milione per rifare qualche chiesa e qualche parrocchia; qualche altro soldo per qualche compagno che sbaglia e così teniamo unito tutto».

cinque punti di riduzione di IRES! Tranne che la base contabile aumenta. E certo, si aumenta la base imponibile

gli interessi passivi o non saranno dedotti, non ci sarà la deduzione forfetaria; chiedo, però, se queste mancate deduzioni di interessi passivi

magari di qualche banca o di qualche grosso gruppo industriale che fa la coda ai banchetti dell'Ulivo per votare, qualche compagno che sicuramente ha qualche banchetta - e ne avete tanti - o forse per il compagno dell'assicurazione, dell'Unipol magari, o per il compagno Montezemolo che ha avuto qualche piccolo beneficio. Ecco, Presidente, i nostri emendamenti vanno nel senso di un taglio.

ma le istituzioni democratiche vanno tollerate. Allora diciamo di cominciare a tagliare dalle consulenze dei Ministeri. Non si può soltanto dichiarare - così come avete fatto nella scorsa finanziaria comma 4 - che ridurrete le tasse, che tutto il nuovo gettito andrà a ridurre le tasse tranne che in certi casi. Capisco le comparsate del presidente Morando e del Governo, grandi vittorie televisive, ma poi vittorie di Pirro nei fatti perché non ci sono state riduzioni di tasse. Quindi, Presidente, cominciamo a tagliare le spese del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia. Cominciamo a ridurre le consulenze. E cosa incominciamo ad aumentare? Incominciamo ad aumentare - per esempio - i trasferimenti all'INPS per i trattamenti delle famiglie. Quando parlate dei privilegi ai parlamentari va bene, ma andate a vedere cosa sta facendo il Ministro dell'agricoltura con gli evasori, con gli SCAU. Chi sono gli SCAU? Sono quelli che, nel mondo dell'agricoltura, non hanno mai pagato una lira!

che, per la massima parte, sono nei vari collegi di quelli che contano nel mondo dell'agricoltura, una volta della passata maggioranza e soprattutto, adesso, della maggioranza attuale. Di quegli evasori non diciamo niente. Primo titolo: «Tagliamo ai parlamentari». Va bene. Ma non si dice nulla su quelli che sono andati a rubare, perché non hanno pagato una lira dei contributi previdenziali in agricoltura:

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge di assestamento per l'esercizio finanziario 2007 riveste ovviamente un carattere propedeutico

- lo dico ai colleghi Baldassarri, Bonfrisco e Polledri - e sicuramente migliore di quello dello scorso anno, e migliore di quello previsto, nonostante la non piena disponibilità - alla data in cui questo provvedimento è stato consegnato, il 30 giugno scorso

Converrebbe adeguare la normativa - mi rivolgo al sottosegretario Sartor - visto che di fatto ogni anno l'assestamento viene discusso e approvato come premessa della sessione di bilancio dell'anno successivo. Forse andrebbe pure rivisitata l'ipotesi l'ipotesi di un ruolo innovativo dell'assestamento mirato anche al controllo degli andamenti di finanza pubblica. Anche quest'anno, infatti, nonostante l'aumento delle entrate tributarie,

il riepilogo della variazione rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2007 evidenzia che sono migliorati i conti, sia in termini di competenza che in termini di cassa. Infatti è migliorato il saldo netto da finanziare, la competenza, è migliorata la cassa. Vorrei fare un riferimento solo numerico: per quanto riguarda l'IRPEF, c'è un aumento di 3.333

all'articolo 15 del decreto di accompagnamento alla finanziaria (un miliardo per il 2007) e li troviamo all'articolo 95, commi 11 e 12, della finanziaria,

per i miglioramenti. Noi vogliamo che siano garantiti i fondi per gli statali. Mi avvio a concludere ponendo soltanto due ultime questioni. È È necessario a nostro avviso, emerge dall'assestamento, modificare la normativa sul 5 per mille che fu definita dal comma 1234 della finanziaria scorsa, prevedendo, lo dico pacatamente, di escludere la scuola non statale ONLUS dai fondi del 5 per mille e anzi, come pur si prevede alla lettera *b)* di quel comma, di impegnare quei fondi a favore dell'università e della ricerca, come da più parti viene chiesto.

Ci preoccupava, lo dissi in quell'occasione, che il terreno della riduzione fiscale venisse limitato al pacchetto casa - ne siamo contenti - e alla semplificazione per le imprese. Ciò si è puntualmente verificato. Al collega Polledri che ci ricorda che l'articolo 1, comma 4, della finanziaria 2007, come è giusto che sia, doveva destinare le entrate tributarie eccedenti, ovviamente se strutturali e permanenti, alla riduzione della pressione fiscale,

che con il decreto e complessivamente con la legge finanziaria possiamo correggere perché, insieme al risanamento, del quale ci complimentiamo per l'azione del Governo, ci sia sempre più equità e sviluppo.

emendamenti. Illustrerò l'emendamento 1.2, dichiarato inammissibile dagli Uffici sulla base di una interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento propone di abrogare il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, il cosiddetto decreto tesoretto, che determina 7 miliardi di spesa dispersa, non coperta finanziariamente, visto che stiamo discutendo oggi l'assestamento di bilancio, e che, di per se stesso, è contrario all'articolo 81 della Costituzione. All'interno di quel decreto ci sono soltanto 900 milioni per aumentare le pensioni minime, 82 centesimi al giorno.

e propone di concentrarli sull'aumento delle pensioni minime non di 82 centesimi al giorno, ma di 150 euro al mese (questo implicherebbe una spesa di 4,3 miliardi) e sull'azzeramento dell'ICI sulla prima casa per tutti (ciò implicherebbe una spesa di 2,3 miliardi), per un totale di 6,6 miliardi, ben al di sotto dei 7 miliardi di spesa dispersi nei vari bilanci ministeriali con la legge n. con la legge n. 127, che, ripeto, convertiva in legge il decreto del 2 luglio, il cosiddetto decreto tesoretto. Concludo, signor Presidente, segnalando la situazione paradossale,

e il decreto che il Governo ha emanato lo scorso giovedì, per un totale di 14 miliardi di euro di spesa, risultano in questo momento totalmente scoperti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Allora mi lasci concludere sottolineando il paradosso: si giudica inammissibile l'emendamento 1.2, nel momento in cui 14 miliardi di euro di spesa pubblica sono palesemente scoperti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e il Governo sta proponendo un assestamento di bilancio - che dovrebbe riguardare soltanto aspetti formali e non sostanziali - di 12,9 miliardi di euro 25.000 miliardi di vecchie lire) di extragettito occultato fino a questo momento, che diventano più 19 miliardi nella Nota di aggiornamento al Documento di e che, secondo i dati del Governo, dovevano essere più 25 miliardi. È un giorno paradossale ma tragico per le Aule del Parlamento quello in cui il Governo palesemente trasgredisce l'articolo 81 della Costituzione e impedisce

le classi deboli, andando a raccontare che date la quattordicesima mensilità ai pensionati e che tenete conto dei non abbienti, senza dire la verità: 82 centesimi al giorno ai pensionati e 42 centesimi al giorno agli indigenti: questo è quanto state approvando mentre il Governo nasconde le cifre! Il paradosso

tecnicamente, e forse giuridicamente, ineccepibile, il paradosso sta in questo, nel momento stesso in cui il Presidente della Repubblica firma due decreti per 14 miliardi di euro palesemente scoperti, contro l'articolo 81 della Costituzione. La ringrazio ancora, signor Presidente, per avermi dato questa ulteriore opportunità. *(Applausi dai Gruppi AN e

il parere sull'emendamento 1.Tab.1.600 del Governo è naturalmente favorevole. Ne abbiamo ampiamente discusso in Commissione e ho riferito qui in Aula, nella seduta della settimana scorsa, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad esprimere un voto assolutamente favorevole a questo emendamento. Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario. Non li menziono singolarmente perché non ve n'è bisogno; trattasi di emendamenti contenenti contenenti appostazioni di maggiori o minori spese che, al di là del merito, tendono a modificare l'effettivo andamento della spesa senza giustificazione alcuna. In realtà, si è voluto

la destinazione del 5 per mille che è stata oggetto di specifico intervento nella legge finanziaria, di cui ci dovremo occupare nei prossimi giorni. Quindi, mi sembra ampiamente superata questa

sugli emendamenti, con l'ovvia eccezione di quello presentato dal Governo, mi unisco al relatore nell'esprimere parere contrario. Come ho avuto modo di dichiarare durante l'illustrazione dell'emendamento governativo, le riallocazioni delle assegnazioni ai singoli Ministeri sono state fatte su proposta dei Ministri al fine di assicurare la massima funzionalità dei Dicasteri stessi; quindi tali correzioni ne impedirebbero, di fatto, la regolare funzionalità, così come ci è stata manifestata dai vari Ministri.

Signor Presidente, credo che raramente i disegni di legge recanti il rendiconto e l'assestamento abbiano destato tanta e tale attenzione,

i motivi di ciò siano sufficientemente noti. Infatti, nonostante la congiuntura economica internazionale estremamente favorevole; nonostante la pace sociale garantita dai sindacati (proprio oggi sul «Corriere della Sera» un articolo riportava in maniera molto chiara che se oggi al Governo, invece dell'attuale Presidente del Consiglio, ci fosse stato Silvio Berlusconi, probabilmente i sindacati sarebbero scesi in piazza per dimostrare contro le nefandezze che questo Governo sta determinando); nonostante la consapevolezza del popolo italiano che ha determinato un incremento delle entrate; nonostante tutti questi fattori favorevoli, state spingendo sostanzialmente il Paese verso il baratro.

a testimoniarlo ci sono anche quei giornali e quegli organi di informazione che a voi sono vicini - come «la Repubblica» - o quelli che a voi si avvicinarono nel corso dell'ultima campagna elettorale, dicendo in maniera chiara come la pensavano riguardo l'espressione di voto e lanciando un segnale molto chiaro alla Nazione. Anche questi organi di informazione sono fortemente critici nei vostri confronti; anche questi organi di informazione si sono resi perfettamente conto che le manovre economiche che state determinando, le scelte politiche che state ponendo in essere, le determinazioni che stanno caratterizzando una maggioranza divisa come non mai non potranno portare risultati probanti ad un'azione politica di Governo che si vorrebbe più incisiva più capace di portare l'Italia a livelli competitivi in Europa e nel mondo; capace, soprattutto, di creare le condizioni e i presupposti per dare un taglio più moderno alla nostra Nazione e al nostro Paese. Quegli organi di informazione sono stati lapidari e precisi nel sintetizzare la vostra situazione, a cominciare dalla legge finanziaria,

una finanziaria per sopravvivere; una manovra - abbiamo già visto i commenti - superficiale, inconsistente, improduttiva, incapace di determinare effetti concreti. Questa è la linea politica che ha caratterizzato la vostra azione di Governo, non solamente negli ultimi mesi, ma da quando avete avuto l'onore di reggere le sorti del Paese. Ebbene, in questa situazione il Senato si accinge a discutere, anzi già discute, del rendiconto e dell'assestamento, da cui emergono alcuni dati significativamente importanti: i conti pubblici sono migliorati grazie alle nuove entrate

una virtuosa azione politica di Governo nella passata legislatura, abbiamo creato le condizioni soprattutto per ripristinare un rapporto di fiducia tra lo Stato, inteso anche come fisco, e il cittadino.

Solamente per questo motivo, e non per una lotta all'elusione e all'evasione che sotto il vostro versante è stata inconsistente, si è avuta la possibilità, quindi, di reperire nuove entrate. al secondo settore, quello delle cosiddette spese stabilizzate, certo, il saldo generale probabilmente potrà aver portato ad una sorta di stabilizzazione e di equilibrio, ma non si dice tutto quando si afferma questo concetto: non si dice, per esempio,

con il risultato finale che questo è un Paese che non investe e che quindi arretra in termini di infrastrutture, di cultura, di quei prodotti finali che lo dovrebbero caratterizzare rispetto agli altri Paesi competitori. Vi è, poi, il tema dei continui tesoretti. Intervengo sull'argomento in questione, sui 900 milioni di euro che sono spuntati da un momento all'altro, dopo che altri tesoretti erano emersi precedentemente. Da questo punto di vista le questioni sono solamente due: o non dobbiamo più credere alla tesi della capacità dell'azione di Governo, che è stata sostenuta a lungo - debbo dire - anche dai Governi e dagli uomini del centro-sinistra, e quindi dovremmo ritenere che abbiamo di fronte dilettanti allo sbaraglio;

con le parole di un autorevole commentatore del «Corriere della Sera» che ha detto che questa finanziaria salva il Governo ma non salva il Paese. Io vorrei correggerlo,

Presidente, noi dovremmo interrogarci sui motivi dell'inconciliabilità e della impossibilità di un rapporto e di qualsiasi forma d'intesa fra l'opposizione e questa maggioranza. La motivazione è soprattutto politica e si fonda sull'esigenza dell'equità sociale, che l'attuale Governo sta del tutto ignorando. Governo lo ammette, un andamento del gettito tributario molto favorevole rispetto alle previsioni. Il bilancio dello Stato può contare su 7 miliardi e mezzo in più. Quindi, i soldi ci sono.

negare una rete adeguata di protezione sociale al cosiddetto lavoro flessibile? Il dramma è tutto qui

Non a caso l'Europa di Prodi fu l'Europa del monetarismo sciagurato: non a caso l'Europa si è sbloccata dopo che Prodi è stato cacciato da Bruxelles, quando ha liberato la sua poltrona. Signori del Governo, dovete prendere atto che avete una sinistra radicale talmente debole e che ha disertato tanto sul fronte dell'equità sociale da da non riuscire nemmeno ad ottenere quelle poche, pochissime misure che erano previste per far sì che il lavoro flessibile fosse accompagnato da una rete di protezione sociale. Non avete nemmeno pensato a sgravare fiscalmente il lavoro dipendente,

il lavoro precario, ad una sinistra di classe, che ha scelto ancora una volta gli interessi della grande finanza e dei banchieri contro gli interessi dei ceti popolari. A qualcuno questo sembrerà un discorso comunista. Ma dietro l'anatema del populismo si nasconde in realtà l'egoismo, l'irresponsabilità, il sordo silenzio,

Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, il senatore Baldassarri ha posto un problema politico rilevante come un macigno: dove sono finiti questi 13 miliardi di euro di cui il Governo ha dato conto nelle settimane scorse come extragettito e che improvvisamente sono scomparsi? È una domanda molto imbarazzante e molto inquietante, anche alla luce del fatto che questi 13 miliardi di euro erano per il 2007. E per il 2007 voglio soltanto citare alcuni dati che testimoniano il fallimento della vostra politica, in particolare sui temi su cui avete vinto la campagna nel 2006. Penso in particolare alla scuola, all'università, alla ricerca. Ebbene, caro ministro Fioroni, lei ha tagliato 200 milioni di euro ai bilanci delle scuole per finanziare la riforma della maturità. Lei ha fatto una controriforma delle superiori a costo zero e poi ha dichiarato di voler rilanciare l'istruzione tecnico-professionale! Lei Lei ha previsto la reintroduzione degli esami a settembre, ma senza adeguati fondi per pagare gli insegnanti perché organizzino dei corsi di sostegno. Forse si ritiene che gli insegnanti debbano lavorare gratis ad agosto? Lei non è stato neanche in grado di provvedere ai fondi sufficienti per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, quando un insegnante si ammalava. È una denuncia della CGIL: mancavano 300 milioni di euro,

Caro ministro Fioroni, lei ha fatto tante belle dichiarazioni, ma poi ha portato il rapporto sull'organico di fatto tra insegnanti di sostegno e studenti da 1 a 138 a 1 a 200: ha quasi dimezzato il numero degli insegnanti di sostegno sull'organico di fatto. Pensate che avete dovuto aspettare l'*Authority* per la concorrenza perché intervenisse denunciando il costo troppo elevato dei libri di testo; non avete neanche provveduto a venire incontro alle esigenze delle famiglie disagiate per consentire che esse possano acquistare gratuitamente i libri di testo. Non avete finanziato il sistema di valutazione delle scuole, non avete consentito la deducibilità delle rette scolastiche, risolvendo dunque quel problema di parità scolastica che potrebbe essere affrontato e risolto senza grossi oneri per lo Stato. Avete soprattutto tagliato risorse imponenti alla scuola italiana. Cari colleghi della 7a Commissione, tutte le settimane, tutti i giorni vi lamentate contro questo Governo per i tagli fatti alla scuola e ora vedo nella bozza di finanziaria che è stata distribuita che addirittura si prevede per il 2008 un taglio di 535 milioni di euro, di 897 milioni di euro per il 2009, di 1.218 milioni di euro per il 2010, di 1.432 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Se questi tagli li avesse fatti il Governo Berlusconi, se li avesse fatti il ministro Moratti, avremmo tutti i sindacati in piazza, avremmo le scuole Oltretutto, vi apprestate anche a replicare la cosiddetta tagliola: mettete la scuola nelle mani del Ministro dell'economia come avete messo l'università nelle mani del Ministro dell'economia. Anche l'università non è stata trattata meglio. Per la prima volta da quando è stato istituito il fondo relativo, i programmi della ricerca per l'innovazione e lo sviluppo sono stati pubblicati a ottobre quando normalmente venivano pubblicati a marzo. Questo vuol dire che il sistema della ricerca italiana, che le università italiane, non hanno avuto a disposizione le risorse per fare ricerca per tutto il 2007, un fatto gravissimo.

Dove stanno, caro ministro Mussi, i soldi per incrementare gli stipendi dei ricercatori? Lei ha detto giustamente che i ricercatori italiani hanno stipendi molto bassi, presto dimenticato che con 1.200 euro al mese questi ricercatori non possono arrivare a fine mese e, quindi, che il mondo dell'università, il mondo della ricerca non è certo attrattivo per i migliori: non ha saputo ottenere risorse adeguate per incrementare significativamente gli stipendi dei ricercatori italiani. Avete persino confermato per il 2008 quella pessima legge Bersani che costringe le università a tagliare sulle spese per il riscaldamento, sui laboratori, sulle biblioteche. Avete finanziato in modo ridicolo, irrisorio, il fondo di finanziamento ordinario per il 2007. Insomma, non siete riusciti a mantenere nessuna delle promesse che avevate fatto in campagna elettorale deludendo il vostro elettorato di riferimento. Andate in qualche scuola, andate in qualche università: i rettori degli atenei italiani hanno persino dichiarato questo Governo non gradito nelle università proprio all'indomani della scorsa finanziaria,

poche decine di milioni di euro su 12.900 milioni in più. E allora, caro ministro Fioroni, la smetta di fare propaganda: ha riempito le pagine dei giornali dicendo che ha reintrodotto lo studio della grammatica e della sintassi nelle scuole italiane. È una balla colossale, perché basta guardare le indicazioni nazionali dell'ex ministro Moratti per vedere che lì quello studio

Caro ministro Fioroni e cara vice ministro Bastico, avete detto che con l'estensione dell'obbligo a 16 anni avete realizzato la più grande riforma della scuola dal 1962: è un'altra balla colossale

Moratti. Anziché riempire le pagine dei giornali con comunicati stampa, con la vostra propaganda, imparate ad essere un poco più seri, cari colleghi. Non lamentatevi più in 7ª Commissione, non approvate più ordini del giorno in cui chiedete al Governo di stanziare risorse significative per la scuola, per l'università e per la ricerca. Cercate di bocciare i provvedimenti che in realtà prendono in giro i vostri elettori e danneggiano il futuro del Paese.

che modifica lo stato di previsione delle entrate e che vorrebbe assestare le entrate in realtà non assesta un bel niente. È la palese dimostrazione che il Governo sta prendendo in giro il Parlamento perché ha ripetutamente modificato la dimensione del gettito. C'è mancanza di chiarezza, venendo meno al principio di trasparenza del bilancio.

di euro. Vogliamo dire le cose con forza, senza infingimenti. Non vengono infatti riportate tutte le entrate nelle cifre reali, non viene spiegata la dinamica di quelle entrate perché si giunge a questo risultato. Onorevole Sottosegretario, in precedenza lei ha fatto riferimento alla caduta, al segno negativo, degli olii minerali, ma non ci ha spiegato la dinamica delle altre componenti delle entrate. [**Presidenza del

un atto di indirizzo unitario, aveva chiesto che fossero aumentate le risorse attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Non lo avete voluto,

Il Governo dovrebbe chiarire l'andamento dell'IVA, che è del 3 per cento sull'anno, e anche l'andamento dell'IRES, che è cresciuta per alcuni soggetti del 400 per cento. Chi sono, onorevole Sottosegretario, questi grandi contribuenti

Ma l'IVA è anche un elemento per valutare attentamente la lotta all'evasione e, in base all'andamento dell'IVA, vediamo che non c'è questa lotta all'evasione di cui si parla. È certo invece che essa deriva da provvedimenti legislativi che voi avete adottato, e non viene invece dal contrasto all' evasione fiscale. Mi domando se il relatore ha letto attentamente la dinamica dell'IVA, la dinamica dei dati mensili, presentati attraverso il bollettino mensile delle entrate tributarie. Credo che non ne abbia fatto una valutazione attenta. Il Governo si era impegnato, in ottemperanza all'articolo 1, comma 4, alla presentazione di una relazione sui risultati del gettito e sulla lotta all'evasione, così non è: dove è questa relazione che doveva essere presentata entro il 30 settembre?

Avete chiuso il 2006 al 43,1. Ciò conferma che le vostre previsioni erano sbagliate, come era sbagliata la *due diligence*, come erano sbagliati i risultati. I dati fiscali al 17 settembre dimostrano che l'IRES è aumentata del 26,3 per cento e del 37,3 nel periodo agosto-settembre. L'IVA è aumentata, come ho detto, del 3,3, quella sulle importazioni è addirittura negativa, segno di una probabile recessione, segno che le imprese non fanno scorte, segno che sono preoccupate dell'andamento e del rapporto euro-dollaro; l'IVA è piatta nel mese di luglio e si presenta debole sugli scambi interni e negativa sulle importazioni. La crescita dell'imposta di registro, che deriva da vostre scelte legislative, con il decreto-legge n. 262, cresce del 25,2 per cento. Questi sono i dati inconfutabili. L'IVA da accertamento e controllo nasce dalla somma di tre voci di gettito realizzate attraverso controllo formale, controllo sostanziale e accertamento con adesione. Gli importi relativi alle prime due componenti non sono disponibili nel *datamart* utilizzato nell'analisi della dinamica relativa di cassa. I diversi princìpi di contabilizzazione non consentono di ottenere dalla somma delle tre componenti esattamente il livello dell'IVA di cassa da accertamento e controllo, anche perché non è stato possibile reperire le somme del controllo formale versate non avvalendosi del modello F24. Il controllo formale ha determinato una crescita della componente a partire dal 2005. Quindi non potete prendere in giro il Parlamento; non potete dire che la lotta all'evasione è vanificata dalle mancate assunzioni alle agenzie fiscali quando avete rifiutato indirizzo del Parlamento per le immissioni in ruolo degli idonei anche laddove la crisi nelle risorse umane era evidente, come in alcune Regioni che formano gran parte del PIL del Paese, come Lombardia, Veneto e Piemonte, preferendo bandire un nuovo concorso con ritardi, costi e minori entrate fiscali. La vostra è oggi una inutile lamentazione. Avete fallito negli obiettivi di politica fiscale e tributaria facendo crescere la pressione fiscale di due punti e mezzo e questo obiettivo viene mantenuto anche per l'anno prossimo, quindi non potete illudere gli italiani. In una recente intervista il sottosegretario Visco ha dichiarato che l'accanimento contro di lui per la questione Speciale è determinato esclusivamente dall'intendimento di ben individuati settori politici, economici, finanziari di eliminare colui che è il fattivo protagonista di una seria lotta all'evasione fiscale. Ma a parte l'affare Speciale, che affronteremo domani, sul quale il Parlamento dovrà fare piena luce e anche tenuto conto delle gravi denunce che sulla vicenda sono state scritte dall'autorità giudiziaria inquirente, sulla pretesa seria lotta all'evasione fiscale occorre fare alcune puntualizzazioni per dimostrare che l'evasione è rimasta di fatto quella endemica di sempre. Premesso che, per aversi recupero di evasione, ci deve essere maggiore presenza di entrate determinate dall'attività di accertamento in uguali condizioni nel tempo di aliquote, basi imponibili e PIL. È ben evidente che se le maggiori entrate derivano da aumenti di aliquote o di basi imponibili si ha soltanto un aumento della pressione fiscale senza recupero di evasione. Ma valga il vero. Dal bollettino delle entrate emanato dal dipartimento per le politiche fiscali risultano accertate per il periodo gennaio-luglio 2007 maggiori entrate pari a 8.140 milioni di euro rispetto all'analogo periodo dell'anno 2006. Tale dato rappresenta il cosiddetto tesoretto inteso come maggiori entrate derivante dal recupero di evasioni fiscali, così come è stato definito dai *mass* *media* su indicazioni della classe politica oggi al Governo. Ma vediamo se le cose stanno così. Subito dopo il suo insediamento il Governo si è dedicato all'inasprimento della pressione fiscale emanando provvedimenti anche d'urgenza che hanno riguardato i diversi settori economici ed impositivi (imposte sulle successioni e donazioni, imposte sui beni d'impresa, IRPEF). Dalle relazioni tecniche risultano maggiori entrate che assommano a 12.519 milioni di euro. Di fatto il recupero di evasione fiscale sarebbe solo di 838 milioni di euro (pari alla differenza tra 8.140 euro accertati e 7.302 come da preventivi del Governo). Elementi più confortanti possono derivare dall'andamento della riscossione tramite ruoli dei tributi diretti e indiretti. Infatti queste sono aumentate nel periodo di una percentuale del 34,2 per cento (anche se in cifra assoluta si tratta di importi modesti). Ma in questo caso si tratta degli effetti di una riforma del servizio di riscossione predisposta dal precedente Governo. Con questi dati ho voluto dimostrare che la lotta all'evasione non è un risultato di questo Governo;

siamo un po' delusi da questa manovra di assestamento, perché purtroppo non lascerà alcuna traccia. Siamo abituati nell'amministrare enti locali, quando usciamo dall'ordinarietà e ci troviamo di fronte ad entrate pesanti e sostanziose per decine di milioni di euro, a porci un problema: abbiamo l'obbligo di lasciare una traccia di questa entrata straordinaria, che deve essere visibile in qualche tipo d'opera o iniziativa, che abbia una funzione. Cosa avrebbe potuto fare a questo punto il Governo? Avrebbe potuto predisporre un piccolo piano di opere pubbliche, un piano straordinario di investimenti e infrastrutturazioni; sappiamo quanto servano nuove infrastrutturazioni in tantissime parti del Paese, proprio per aiutare un'economia pro futuro, che oggi è strozzata in gran parte anche dall'incapacità di competere

ammortizzare una bella fetta di debito pubblico, che poi sappiamo essere la nostra bestia nera; ogni anno ci confrontiamo con i parametri

Si sarebbe potuto fare altro. Abbiamo un inverno, colleghi, che per chi abita nelle Regioni del Settentrione si prospetta di non tranquillo inizio. Abbiamo due dati importanti. L'*Authority* per l'energia e l'ENEL ci dicono che non abbiamo le risorse necessarie per affrontare quella crisi energetica che ogni ogni stagione invernale ci prospetta. Non ci sono soldi, oltre ad esserci un Ministro che blocca tutte le iniziative. Il Governo avrebbe potuto tranquillizzare gli italiani annunciando un massiccio intervento per

Vivaddio, si sbloccasse anche il grande tabù del nucleare in Italia: un nucleare pulito, un nucleare di quarta generazione, un nucleare al quale ci rivolgiamo ogni giorno per acquistare energia facendo finta di essere a posto, perché in questo Paese un *referendum* ha sancito che sul nucleare non si potrà più continuare. Si sarebbe potuta fare un'altra grandissima operazione, cara alla sinistra, un'opera di grande redistribuzione. Ci sono famiglie, lavoratori, pensionati che non ce la fanno più a chiudere il bilancio mensile Ebbene, una politica seria dei redditi (lì si sarebbe dovuto fare un vero investimento), una politica quasi keynesiana potrebbe mettere in moto una seconda economia derivata da consumi che oggi non ci sono e che sarebbero fortemente messi in moto da capacità e da risorse nuove da poter destinare in qualche modo - grazie a studi del Governo - a favore di famiglie, lavoratori e pensionati. Nemmeno questo si è fatto.

l'ennesimo ricatto di una piccola componente di questo Parlamento, di una piccola componente della sinistra che -

anni. L'Italia va in controtendenza e questo Governo - lo abbiamo già capito - ha ceduto all'ennesimo ricatto e scorporerà questa parte non da questa manovra e probabilmente nemmeno dalla finanziaria; ritarderà il *redde rationem* e spera di sopravvivere sopravvivere ancora un po'. Ebbene, nulla di positivo e di concreto sarebbe potuto rimanere in termini di investimenti, di infrastrutturazioni, di rilancio dei consumi, di di riduzione della pressione fiscale riducendo il debito; potendo ridurre il costo dell'indebitamento, si sarebbe potuta fare una politica di riduzione dell'imposizione fiscale. Bene, si è persa l'ennesima occasione.

a giochi di prestigio contabili. L'abbiamo visto l'anno scorso, quando era evidente a tutti, da numeri assolutamente incontrovertibili, che c'erano quasi 40 miliardi di maggiori entrate fiscali nel corso dell'anno, maturate per la maggior parte nel periodo di Governo della Casa delle

Si è fatta una finanziaria, come tutti ricordiamo e come tutti quotidianamente possiamo constatare, di lacrime e sangue, assolutamente inutile, perché sostanzialmente ha tassato chi già pagava le tasse, non ha trovato alcun evasore e, soprattutto, non ha

in quest'Aula è stati in grado di chiarirlo. Evidentemente, visto non si possono nascondere fisicamente, le maggiori, drammatiche uscite in aumento aumento della spesa corrente pubblica sono state in qualche modo mascherate dal consumo nascosto di quelle maggiori entrate. Oggi siamo qui a fare e a dire le stesse cose; stiamo infatti assistendo anche quest'anno ad un maggior gettito

Il primo ministro Prodi, il ministro Padoa-Schioppa e gli altri personaggi principali della compagine governativa vanno ogni giorno in televisione a sproloquiare sulla situazione economica incredibilmente e velocissimamente migliorata da questa maggioranza, sparando numeri del lotto o comunque numeri che solo loro conoscono, ma che nessun istituto internazionale (o anche semplicemente gente normale e comune e le stesse famiglie che quotidianamente fanno fatica a vivere) riesce a individuare

i conti pubblici italiani sono stati finalmente messi in ordine. Questa è la parola magica che ogni volta viene tirata fuori. Vorrei capire cosa si intenda con l'espressione «aver messo in ordine i conti pubblici», dal momento che l'indebitamento complessivo, quindi il debito dello Stato, fisicamente è aumentato anche quest'anno, esattamente come gli anni scorsi, forse anche un pochino di più, e vedremo poi quale sarà il numero finale. Lo sfondamento della spesa corrente sul PIL, quindi il *deficit* di bilancio annuale, varia amabilmente dall'1,5 al 4 per cento a seconda delle trasmissioni televisive che si seguano o degli articoli di giornale che si leggano. La pressione fiscale è drammaticamente aumentata, sia sulle famiglie che sulle categorie produttive, ma sul punto

in cui proprio le classi più deboli, le persone che prendono 1.100 o 1.200 euro al mese, che hanno la famiglia da mantenere, denunciavano un incremento della tassazione. Questo è il risultato di tutti gli artifici contabili fatti in finanziaria, dove sono stati fatti giochi di prestigio sulle aliquote; si è intervenuti sulle detrazioni e sulle deduzioni: il «*bonus* bebè» è stato tirato via; il famoso assegno che, secondo Prodi, doveva accompagnarci

avete introdotto l'IRAP. Guarda caso, in un Paese che ha il problema della scarsa capitalizzazione delle imprese e ai tempi aveva un problema di forte disoccupazione, avete introdotto una tassa che tassa gli interessi passivi che pagano le imprese ed il costo del lavoro.

gli evasori. Mi permetto una annotazione: chi ha una partita IVA, un'attività in regola, ha comunque un bilancio che un commercialista esterno gli prepara; non appartiene esattamente al mondo degli evasori, che sono quelli che non hanno né commercialista, né bilancio e magari neanche partita IVA, ma lavorano lo stesso.

costano centinaia di euro ogni mese di commercialista, per burocrazia inutile. Mi piacerebbe sapere quanta evasione avete recuperato con l'introduzione dell'elenco clienti-fornitori. Ve lo dico io: zero! Avete solo fatto pagare soldi che, magari, sarebbero stati impiegati nell'acquisto di una macchina utensile, nella costruzione di un capannone, nell'introduzione di una automazione e che

di persone a tempo determinato, facendole diventare a tempo indeterminato nello Stato; ne avete assunti altri 60.000-70.000 qualche mese fa nella scuola. Avete in definitiva portato oltre i 5 milioni i dipendenti pubblici in questo Paese, a fronte di neanche 23 che lavorano.

che siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti, quindi nella fase che precede quella più propriamente dedicata alle dichiarazioni di voto sul primo degli emendamenti e al voto. Presidente, intervenendo per avere un chiarimento, però, mi consenta, anche per dissentire da questa comunicazione. Come risulta dal resoconto stenografico, seppure in bozza, il Presidente dell'Assemblea, in occasione di una richiesta di intervento del senatore Novi, ha dichiarato chiusa la fase dell'illustrazione e ha detto al senatore Novi che gli avrebbe dato la parola subito dopo per dichiarazione di voto. A quel punto, come propriamente prevede il Regolamento, il Presidente ha dato la parola al relatore esprimesse il parere sugli emendamenti. Subito dopo, ha chiesto il parere del Governo, che è stato conforme, e quindi ha cominciato a dare la parola per dichiarazione di voto.

Siccome ho percepito che si trattasse di un *lapsus* formale, mi sono avvicinato al banco della Presidenza e gli autorevoli rappresentanti del Servizio dell'Assemblea mi hanno confermato che appunto di *lapsus* si trattava. Ora, Presidente, vorrei capire se siamo tornati nell'ambito del Regolamento e si stanno svolgendo le dichiarazioni di voto sul primo degli emendamenti oppure se, come accade da un po' di tempo (dal mio punto di vista, da un anno e qualche mese), ancora una volta abbiamo abbiamo affiancato alle previsioni del nostro Regolamento, alla consuetudine e alla prassi, anche qualche novità. Vorrei almeno chiedere che ciò non costituisca un precedente, altrimenti se ogni volta che relatore e Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti abbiamo la possibilità di riprenderne la discussione e l'illustrazione, lei comprenderà

a ciò di cui mi è stata data informazione, mi risulta, e il Regolamento lo prevede, che la discussione degli articoli inizi con l'illustrazione degli emendamenti. Successivamente ad essa, e prima che vi siano i pronunciamenti del relatore e del Governo, c'è la discussione sull'articolo. L'unica anomalia rispetto a ciò è che, a conclusione dell'illustrazione degli emendamenti, è stata data la parola al relatore e al Governo, dopodiché si è aperta la discussione sull'articolo.

Questa interpretazione degli uffici, anzi, si ritrova rispetto ad un'evenienza connotata da un'interpretazione già ristretta e non penso possa essere ristretta ancora di più, perché si tratterebbe di una compressione del nostro diritto.

che, tutto sommato, sia stato un bene commettere questo piccolo strappo regolamentare perché ci ha permesso, se non altro, di comprendere le ragioni per le quali il relatore e il Governo si sono espressi in senso contrario agli emendamenti

perché l'Esecutivo assume che questa verifica delle maggiori entrate deriverebbe, in sostanza, da attitudini comportamentali diverse dei contribuenti in relazione alla nota vicenda dell'IVA automobili. Come mai questa diversa attitudine dei contribuenti si riflette oggi sull'IRES, mentre il Governo stesso in sede di Commissione aveva assunto che le variazioni che aveva proposto relativamente all'IRE derivavano proprio dalla cosiddetta questione IVA auto? o tale questione riguarda entrambe le imposte (e pertanto sarebbe stato opportuno ottenere delle spiegazioni più circostanziate), oppure ‑ cosa che temo - in qualche modo il Governo è andato per approssimazioni successive, variando il livello complessivo delle entrate e scoprendo ogni piè sospinto un nuovo tesoretto, senza in realtà avere una chiara motivazione delle modifiche che ha apportato al totale delle entrate, né una chiara spiegazione logica di quanto è avvenuto. Se così non è - e temo che per certi aspetti così non sia - ne possiamo dedurre che la consistenza, non dico esatta all'euro ma per per quanto è possibile fare, non corrisponda alla realtà, ma sia sostanzialmente un ottativo da parte del Governo o un'approssimazione che nel corso dell'anno potrà essere smentita dagli eventi. Mi riferisco in particolare anche al fatto che il Governo stesso, nella relazione previsionale e programmatica presentata in questi giorni al Parlamento e al Paese, ammette che per certi aspetti possa realizzarsi un diverso andamento dell'economia, con riferimento agli effetti della crisi del *subprime*, che, come tutti sanno, ha colpito i mercati immobiliari mondiali. Se così fosse, allora mi domando come mai il Governo abbia presentato una variazione che non sarà consistentissima, ma che, combinata con quella che era già contenuta nel primo emendamento approvato in sede di Commissione bilancio in materia di entrate, fa sì che la variazione complessiva delle entrate sia assai consistente. L'emendamento presentato all'Aula aumenta in costanza di un andamento dell'economia e di possibili riflessi sulle entrate non del tutto chiari e probabilmente non così favorevoli nell'ultima parte dell'anno, come dimostra anche l'andamento della produzione industriale

a meno che con esso non si sia voluto non fare un'operazione di verità sulle entrate - cosa che sarebbe la specifica attitudine degli emendamenti all'assestamento per quanto riguarda principalmente le entrate - ma compiere un'operazione esclusivamente finalizzata a garantire copertura finanziaria ad una serie di spese. Come sostengono i giallisti, due indizi fanno una prova: uno è questo emendamento; il secondo è il decreto-legge che accompagna la finanziaria, che copre una serie di spese che francamente potevano essere evitate. Forse queste spese servono nel vano e ultimo tentativo di tenere insieme, per via monetaria e finanziaria, una

Non è piovuto dal cielo, signor Presidente: sono soldi dei contribuenti e qualunque persona di buonsenso farebbe bene a restituirli ai contribuenti piuttosto che pensare di spenderli per altri motivi. Detto questo, è significativamente preoccupante il fatto che siano stati definiti questi tesoretti e che essi vengano utilizzati per coprire il decreto‑legge che accompagna la finanziaria. In sostanza, l'impressione che si ha è che, anziché essere calibrati esattamente sul livello presunto delle entrate (che, come mi sono permesso di dire, non è assolutamente certo, soprattutto per quanto potrà succedere negli ultimi mesi dell'anno), siano esattamente calibrati rispetto alle necessità finanziarie di coprire questo decreto di spesa. In sostanza, il Governo non ha compiuto un'operazione di verità sulle entrate, ma si è limitato a precostituire un meccanismo di copertura. Tra l'altro, se volessimo veramente ragionare in termini di copertura, credo che un attento esame, non solo del Parlamento, ma anche della suprema magistratura, quella che

signor Presidente, come ella sa e come sanno benissimo tutti i colleghi, è assolutamente contrario alla legge di contabilità, non solo in generale, ma tanto più nello specifico, in quanto entrate *una tantum*, probabilmente non ripetibili nel corso degli anni (di cui quindi non abbiamo la sicurezza che esista un futuro di stabilità), servono a finanziare spese che invece rimarranno fisse. Si tratta di un meccanismo di copertura assolutamente non condivisibile e censurabile, che quindi non può essere utilizzabile; ciò nonostante il Governo l'ha utilizzato e - ahimè - temo che l'abbia fatto precostituendosi le entrate con appostazioni contabili su questo disegno di legge di assestamento. Questo per quanto riguarda le entrate. Per quanto concerne gli emendamenti che modificano alcune unità previsionali di base relative alla spesa, sono rimasto francamente stupito del fatto che il relatore abbia espresso un diniego assoluto senza motivarlo e che il Governo abbia assunto il fatto che le modifiche contenute nell'assestamento derivano dalle necessità gestorie dei Ministeri. Allora, signor Presidente, su alcuni settori di spesa, già illustrati dai colleghi, era forse opportuno concentrare di più la spesa per risolvere problemi reali e seri.

il non invidiabile primato storico di avere il maggior numero di Ministri e Sottosegretari della storia repubblicana. Se volessimo sinceramente guardare a questo settore, forse dovremmo intervenire da subito diminuendo il numero dei Ministri e dei Sottosegretari, piuttosto che aumentarlo ancora una volta.

l'impalcatura del bilancio, e il sottosegretario Sartor lo sa bene, si imposta in funzione della spesa storica o dell'entrata storica e in funzione del divenire della stessa. All'epoca in cui le entrate dello Stato davano già segni di lievitazione notevole eravamo in tempo per contemplare l'eventuale maggiore entrata

si sarebbe comportato così, posto che le entrate, per qualsivoglia motivo (ma noi lo conosciamo bene), hanno lievitato in funzione dei provvedimenti che il Governo di centro-destra aveva a suo tempo varato, determinando

avrebbe dovuto postulare una contrazione della pressione fiscale, posto che la finalità statuale e quella del governante non è quella di torchiare per avere maggiori entrate e provocare maggiori spese, quanto quella di provocare entrate in funzione del fabbisogno finanziario per il funzionamento dello Stato. Vero è che una visione collettivistica dello Stato, quale quella di questo Governo, fa sì che sia virtuoso provocare un incremento delle entrate per provocare un incremento delle spese. Poi, con gli emendamenti dei quali è dato avere notizia oggi e dei quali stiamo discutendo, è possibile evidentemente decidere come trattare questo popolo, che non è più il popolo dei cittadini e perciò non è più governato democraticamente. È un popolo che diventa popolo di sudditi e, quindi, subisce prima la torchiatura e poi l'erogazione in funzione del desiderio di provocare una *captatio benevolentiae* a fini elettorali.

e abbiamo l'obbligo di far sapere al popolo italiano che voi avete preteso più entrate di quante potevate chiedere per il normale funzionamento dello Stato! Voi avete determinato il contribuente a dare, vuoi come famiglia, vuoi come imprenditore, più di quanto doveva e poteva dare per far funzionare lo Stato. Voi oggi, con questa impalcatura contabile, orientate il flusso, che è frutto di lavoro e di sacrificio della famiglia e dell'impresa, per una spesa per buona parte corrente, per una parte che non produce, dopo averla sopportata, nessun effetto favorevole per l'avvenire. Avete contratto la spesa per investimento ancora una volta e avete orientato il sacrificio della gente per finanziare spese che devono provocare sola *captatio benevolentiae*. Ma il popolo italiano ha capito perfettamente che per essere governato ha bisogno di chi chiede quanto meno possibile come contribuzione e che spende possibilmente nella direzione di porre le premesse per provocare una redditività futura maggiore di quella che si è verificata in passato. Voi dilapidate anche quello che la provvidenza

tende a reagire con un certo nervosismo, anche perché il tesoro, nell'immaginario collettivo è associato ai pirati e si ha la sensazione, infatti, di essere stati depredati come se il Governo fosse, appunto, composto da pirati. Ma questa è una notazione solo polemica

continua a sostenere la tesi, totalmente destituita da ogni fondamento, che l'incremento delle entrate sia frutto della lotta all'evasione fiscale. Perché questa tesi è destituita di ogni fondamento? Non certo perché

Supponiamo che fosse vero che l'attività di contrasto all'evasione fiscale condotta dall'amministrazione finanziaria dello Stato abbia subito un impulso così significativo come quello che il Governo vuol farci credere. Non è vero: chiunque conosce la situazione reale, i dati che vengono presentati dalla Guardia di finanza sa che l'attività di accertamento non è né calata né aumentata negli ultimi anni, ma si mantiene nel suo *standard*, ma supponiamo pure che questa attività sia aumentata in una maniera straordinaria, grazie all'impulso dato da questo Governo. Orbene, chiunque conosca le regole del procedimento e del contenzioso tributario sa benissimo che anche se oggi noi iniziassimo un contrasto all'evasione con milioni di finanzieri alla caccia dei milioni di evasori non vedremmo il denaro in cassa prima di 10 o 12 anni, perché questo è il tempo che occorre tra il momento in cui si fa un accertamento e il momento in cui la giustizia tributaria dirime la controversia con il contribuente ed eventualmente lo condanna al pagamento. E solo a quel punto si ha l'esazione della somma. Allora, signor Presidente, non si può raccontare agli italiani - i quali queste cose non le sanno per loro fortuna perché non incappano tutti i giorni nella giustizia tributaria, essendo circondati dall'ingiustizia tributaria di un Paese che li costringe a pagare il 45 per cento quando fanno un lavoro dipendente qualunque, una tassazione che nessun altro Paese al mondo mette - la bugia della lotta all'evasione per giustificare il fatto che il Governo invece in ogni piega della tassazione ha aumentato le aliquote, ha aumentato la pressione.

di crescita che c'è stato, è inevitabile che le entrate aumentino, è una deriva che è stata in qualche misura favorita dal fatto che un altro Governo ed un'altra maggioranza hanno rovesciato la prospettiva sull'evasione e forse hanno consentito a questo Governo e a questa maggioranza di raccogliere qualche frutto. Vede, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il vero contrasto all'evasione fiscale in tempi della nostra generazione e non della prossima, non lo si fa schierando milioni di agenti di polizia tributaria o facendo la faccia feroce, o dicendo che si fa la lotta all'evasione fiscale, perché queste sono parole che fanno ridere soprattutto coloro che al Fisco sono sconosciuti, cioè gli evasori totali, che se la ridono della grossa. La vera lotta all'evasione fiscale la si la si conduce riducendo le aliquote e rendendo vantaggioso a chi fino ad oggi non ha aderito al patto fiscale, per qualunque motivo egli lo abbia fatto - e non sta a noi moraleggiare sul motivo per cui lo ha fatto se abbiamo interesse che rientri nella legalità fiscale - consentendo percorsi di rientro nella legalità fiscale attraverso i tanto famigerati condoni, che invece sono misure di sana politica fiscale quando si riforma il sistema e si abbassano le aliquote, perché si consente di ripartire da zero avendo riconosciuto che il precedente sistema era iniquo e provocava danni innanzitutto alle entrate e all'Erario. alle entrate e all'Erario. Questo è quello che è successo negli ultimi tre anni, forse direi in quattro su cinque anni del Governo Berlusconi, a partire dal tanto vituperato scudo fiscale che ha fatto rientrare in Italia i capitali che adesso ritornano ad uscire quanto più velocemente possono, perché anche su quella misura è gravata durante la campagna elettorale la minaccia della sinistra radicale di ritornare su quei contribuenti per dargli una stangata aggiuntiva perché non era stata sufficiente energica l'aliquota posta dal Governo - e da allora fino alla fine della legislatura c'è stato un progressivo rientro nella legalità fiscale favorito dal Governo e dallo Stato. È questo che sta all'origine dell'aumento delle entrate tributarie. Non è un caso, signor rappresentante del Governo, signor Presidente, che questo flusso positivo stia dando adesso una controtendenza. È sufficiente correlare le curve della pressione fiscale, della sua discesa e del suo incremento, con le curve delle entrate allineandole sui periodi di imposta per vedere come la diminuzione attesa delle entrate fiscali è il frutto dell'inasprimento e della tassazione sopra ogni dimensione provocata dalla prima finanziaria del Governo in carica.

perché i più colpiti sono quei lavoratori dipendenti di cui si afferma invece la volontà di difenderne il potere di acquisto, e sono stati martoriati dalle tasse. L'altro giorno, signor Presidente, ho parlato con un insegnante di scuola media superiore, che occasionalmente collabora alla stesura di alcuni libri di testo e che per una marginale collaborazione, pagata al lordo 4.000 euro, ha visto gravare un'imposizione fiscale del 45 per cento su quella parte marginale di reddito. Ed è un insegnante di scuola media superiore con una normale anzianità ed un normale - anzi un normalmente indecoroso - stipendio. Eppure tutto questo lo classificate, signor rappresentante del Governo, come lotta all'evasione e alla grande evasione, come riequilibrio sociale, come misura a favore dei poveri e contro i vituperati ricchi. Conoscete la verità dei vostri conti? La verità dei vostri conti è che gli evasori totali crescono e, per parte mia, mi sento di dire che, proprio perché la vostra politica fiscale è così, non avrete altro che questo risultato: crescerà sempre di più l'evasione, anche quella marginale, e anche quell'insegnante di cui parlavo prima cercherà di farsi pagare in nero e, per quanto mi riguarda, dico che farebbe bene. *(Applausi

Signor Presidente, devo dire che guardando l'insieme dei provvedimenti che in questo periodo sono in discussione nelle Commissioni e in Aula,

verso nuove elezioni che metteranno fine a questa esperienza che è stata decisamente infelice. Perché dico questo? Perché vedo una serie di misure, di tentativi di misure, che sono chiaramente dettati dalla disperazione e dal tentativo di raddrizzare un pochino la barca che sta affondando o quantomeno di creare qualche scialuppa di salvataggio per di salvataggio per la numerosissima coalizione, la numerosissima aggregazione di partiti, di Ministri, di Vice ministri e di Sottosegretari che questa barca stanno molto malgovernando. Uno dei sintomi lo troviamo in questo legge di assestamento del bilancio. Siamo stati accusati, il precedente Governo della Casa delle Libertà, il Governo Berlusconi, è stato accusato di aver creato paurosi buchi di bilancio. una balla assoluta, usata prima in campagna elettorale e poi come pretesto per la stangata della scorsa manovra finanziaria, dello scorso decreto Bersani e di altre misure vessatorie nei confronti dei contribuenti.

al Governo Berlusconi la colpa delle tasse che l'attuale Governo vuole imporre, per motivi ideologici e allo scopo di finanziare una spesa pubblica che si vuole incrementare (altro che tenere sotto controllo). controllo). Il tentativo è dunque quello di dare la colpa alla gestione precedente. L'idea era poi di andare avanti e, dopo un periodo credibile di almeno due o tre anni, scoprire improvvise nuove entrate ed usare questo denaro non già per ridurre le tasse ai cittadini, se non in modo estremamente marginale, ma per fare qualche regalia elettorale. Questo piano si è però dimostrato fallimentare. Intanto gli italiani hanno capito benissimo che chi aumenta le tasse ha la responsabilità di farlo e non può dare la colpa a chi ha lasciato i conti in ordine e a chi, durante il periodo in cui ha governato, le ha diminuite. In secondo luogo il piano è fallito perché il consenso dell'attuale maggioranza è talmente basso nel Paese e la situazione politica nel suo insieme è talmente compromessa che questo piano, che aveva bisogno di almeno due o tre anni per avere una sua realizzabilità, ha dovuto essere anticipato e dunque, appena finito di dire che c'era il buco spaventoso lasciato dal Governo Berlusconi, si è dovuto dire che al posto del buco c'era il tesoretto A, il tesoretto B e tanti altri tesoretti. tesoretti, per altro, il contribuente non ha visto traccia, perché il tesoretto l'ha tirato fuori lui, l'hanno tirato fuori i contribuenti, dalle proprie tasche per finanziare la spesa pubblica in aumento. aumento. Il fatto di dover comprimere così tanto i tempi di questa commedia è chiaro sintomo che la commedia, grazie al Cielo, sta per finire, ma ci sono altri elementi che indicano che siamo all'atto finale di questa triste commedia e sono per esempio i provvedimenti che vediamo nella legge finanziaria che è stata licenziata dal Governo e che inizierà il suo *iter* qui al Senato, che contiene delle misure di finanziamento, di clientela e delle misure che che vengono apparentemente incontro ai redditi più bassi, che alla fine si concretizzano nella riduzione della bellezza di 40 centesimi al giorno di imposte per famiglie che si trovano in situazioni particolari. A fronte di questo, abbiamo degli atti che dovrei dire inconsulti: abbiamo nella finanziaria - questo indica proprio che siamo a fine corsa - una radicale radicale riforma della strutturazione delle amministrazioni locali, abbiamo la ristrutturazione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e delle Comunità montane contenute nella finanziaria, per questo Governo le amministrazioni locali non sono un fatto istituzionale che dunque dovrebbe essere riformato secondo il normale *iter* che si deve seguire per le riforme istituzionali, e cioè nelle Commissioni competenti, con un provvedimento a sé stante: sono considerate solo un costo e dunque essendo solo un costo vengono trattate dalla finanziaria. Ma allora, se sono un costo, sarebbe più coerente sopprimerle del tutto, si mettono tanti amministratori unici come quello che Veltroni vorrebbe mettere alla RAI,

Chi ha un'idea a quanto ammontino le retribuzioni dei Consiglieri comunali dei Comuni dai 3.000 ai 10.000 abitanti ha idea di quanto si risparmi con questa misura questa misura e la misura infatti di questo risparmio è contenuta nella relazione tecnica allegata agli articoli della finanziaria, e cioè zero, senza contare che molto spesso gli amministratori di questi piccoli Comuni sono persone che finiscono per fare volontariamente attività per le quali altrimenti bisognerebbe assumere qualcuno e non mi riferisco ovviamente all'attività amministrativa, ma a lavori inerenti il funzionamento dei servizi che il che il Comune si sforza di dare ai cittadini. Se poi nell'ambito di questi amministratori comunali ci sono dei disonesti, evidentemente se ce ne sono di meno non vuol dire che saranno meno disonesti; questo indica proprio un gesto di disperazione, cioè chi governa, che dovrebbe avere il compito di risanare quello che c'è da risanare, di riformare quello che c'è da riformare, di dare una risposta ai problemi reali del Paese, non riuscendoci e non riuscendoci in particolare in quei settori in cui più ha insistito durante la campagna elettorale e nella prima parte del Governo, non riesce a dare risposte. Mi riferisco al problema del precariato, su cui si è fatto un grande *battage* in campagna elettorale, falsificando la realtà e cioè e cioè attribuendo al Governo Berlusconi l'introduzione del precariato, che semmai è stato reso più regolamentato, con maggiori garanzie per il lavoro, perché sappiamo bene che questa tipologia di contratti fu varata soprattutto nel 1998 e dunque sotto il precedente Governo di centro-sinistra, su questo ha molto puntato il centro-sinistra in campagna elettorale, facendo credere che una volta mandato via il Governo Berlusconi e la Casa delle Libertà, sarebbe cessato il precariato, tutti sarebbero stati assunti stabilmente, a tempo indeterminato, e così via. Ebbene, siccome assolutamente nulla è successo di questo genere

ciò dovrebbe incentivare il passaggio a tempo indeterminato, ma è chiaro che può essere avvenuto in un numero così ridotto di casi che non è certo paragonabile con un numero certamente maggiore di casi in cui si è ritornati si è ritornati dal precariato al lavoro nero, che indubbiamente non è un progresso. Allora, quando di fronte a tutto questo, di fronte alle promesse fatte, l'unica cosa che riesce a realizzare questo medico che dovrebbe essere il Governo - il medico dei mali del Paese quale si era proposto - è fingere di fingere di abbassare la propria parcella, riducendo il numero dei consiglieri comunali, anche dei piccoli Comuni, ebbene, questo è un segno di resa e di disperazione che rappresenta una buona notizia per il Paese, perché i danni che questo Governo ha fatto e che deriverebbero dall'approvazione dei parecchi provvedimenti che in qualche modo, molto a rilento, vanno avanti nelle Camere, sarebbero troppo pesanti perché questo Paese li possa sopportare. Speriamo che l'ultimo atto della commedia finisca presto e che si vada a nuove elezioni. *(Applausi dal volevo fare una proposta all'Aula rispetto ad una richiesta che mi è stata formulata dal Governo. Trovo che fino a questo punto ci siamo sufficientemente assestati; abbiamo una richiesta da parte del vice ministro Danieli perché possa essere

e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

della ratifica, o meglio, del rinnovo di un Accordo tra l'Unione Europea nel suo insieme e i Paesi africani. È pertanto qualcosa sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, anche per l'impegno straordinario:

certamente più urgente e avente una scadenza definita. Vorrei però sottolineare che da questa sera - e non è la prima sera - la Repubblica italiana ha due provvedimenti, una legge e un decreto, completamente scoperti, in base all'articolo 81 della Costituzione, per oltre 14 miliardi di euro. La pregherei, signor Presidente, di far rilevare questo anche alla Presidenza della Repubblica.

con i senatori Del Roio, Mele e Cossutta riguarda una questione molto importante collegata al disegno di legge che stiamo discutendo. Mi riferisco alla necessità di assicurare che gli Accordi di partenariato economico, ovverosia gli accordi commerciali che l'Unione Europea sta negoziando con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, siano improntati a criteri di equità, giustizia economica e sociale e reciprocità. Il problema fondamentale è che ad oggi, per come vengono impostati tali accordi, si corre il rischio che i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico debbano accettare condizioni che rischiano di contraddire alcuni degli obiettivi fondamentali dell'Accordo di Cotonou, che sono principalmente la lotta alla esclusione sociale e la lotta alla povertà. Quindi, anche sulla scorta delle grandi mobilitazioni svolte la settimana scorsa a livello internazionale sui negoziati EPA, chiediamo che il Governo italiano possa assicurare una maggiore valutazione rispetto alle ricadute di sviluppo di questi accordi,

presidente del Burkina Faso, il quale mise al centro del suo impegno proprio il tema della giustizia economica nei confronti dell'Africa, un impegno che non possiamo assolutamente dimenticare. Dobbiamo poi sottolineare anche come l'Unione Europea rischi di venire meno a tali impegni se non garantirà che negli accordi commerciali verso quei Paesi venga messa al centro la lotta alla povertà e non la liberalizzazione negli scambi commerciali e dei servizi. Colleghi, non so se è noto a tutti quelli che amabilmente stanno chiacchierando nell'emiciclo che stiamo trattando un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale. Non vorrei minacciarvi di tornare a trattare l'assestamento se non si libera subito l'emiciclo.

Per quanto riguarda però l'ordine del giorno G1, che apprezziamo per lo spirito, ci asterremo perché stiamo chiedendo al Governo un impegno che credo difficilmente potrà potrà essere mantenuto. Se è un auspicio ed un impegno ad operare affinché questo avvenga potremo convenire. Sull'ordine del giorno francamente devo dire

Colleghi, volevo fornire all'Assemblea una comunicazione e un chiarimento. Quanto alla comunicazione, riflettendo bene, anche nell'interesse dell'Assemblea, avendo noi già per un pomeriggio la diretta televisiva per il dibattito sul problema vice ministro Visco-Guardia di finanza con l'intervento del Ministro dell'economia,

Se lei ci convocherà, ci presenteremo, ma ritengo che questo dibattito sia stato utile ed interessante e non credo di condividere le eccessive preoccupazioni della collega Finocchiaro perché abbiamo tempo